"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

l'elemento tragico da cui parte il disegno di legge in discussione è la tragedia avvenuta il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. Il naufragio di una delle famigerate carrette del mare portò alla morte ben 368 persone, compresi anziani, donne e bambini. All'indomani di quella tragedia si costituì il Comitato 3 ottobre, una ONLUS che ha lavorato perché quella triste data, attraverso l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, potesse diventare non solo un momento di ricordo e commemorazione delle vittime, ma innanzitutto l'occasione per rafforzare, attraverso il principio di solidarietà, quell'identità europea che è parsa del tutto smarrita negli eventi degli ultimi anni, mesi e settimane. In questo In questo momento mi preme ringraziare il Comitato 3 ottobre, che ha voluto fortemente il ricordo di questa data tragica e tutti i cittadini di Lampedusa, con in testa il sindaco Nicolini, che si sono tanto prodigati per soccorrere le vittime dei tanti naufragi che si sono susseguiti negli ultimi anni nel Mediterraneo. Il 3 ottobre è, quindi, una data simbolica importantissima, ma le morti legate ai trasferimenti di migliaia di persone in Europa sono state numerose anche prima e dopo

signora Presidente. Dicevo che il 3 ottobre è da considerare una data simbolica molto importante, ma mi preme anche ricordare che le morti legate ai trasferimenti di migliaia di persone in Europa sono state numerose anche prima e dopo quel 3 ottobre 2013, che resta comunque una data chiave nella storia dell'Europa e dell'immigrazione. Dopo quella tragedia, che sembrò sconvolgere le coscienze di mezza Europa, il Governo Letta decise di avviare l'operazione Mare nostrum, che avrebbe poi chiuso il 1° novembre 2014. operazione aveva due obiettivi fondamentali: garantire la ricerca e il salvataggio nelle acque internazionali dei migranti e assicurare alla giustizia trafficanti e scafisti. un impegno oneroso (nove milioni di euro al mese) e di un'esperienza finita nel mirino delle polemiche, perché accusata di aver moltiplicato il numero dei disperati salpati dai porti del Mediterraneo meridionale, attirati dalla certezza di essere soccorsi in mare. Mare nostrum ha salvato 150.000 persone e dopo la sua chiusura gli arrivi sulle nostre coste meridionali sono aumentati insieme alle richieste di asilo. Quindi, Mare nostrum non era la calamita dei disperati. Le calamite e le cause andavano ricercate altrove. Ma ancora una volta, a imprimere una svolta al corso degli eventi, dopo le tante polemiche, è stata la cronaca: il 18 aprile 2015, nel naufragio di un barcone proveniente dalla Libia morirono oltre 700 persone, forse 900. Due giorni dopo, un vertice congiunto dei Ministri degli esteri e degli interni dell'Unione europea partorì un piano in dieci punti che prevedeva il rafforzamento delle operazioni nel Mediterraneo, lo sforzo sistematico per catturare e distruggere i barconi, asylum support office (EASO) per sveltire le pratiche delle richieste di asilo, lo studio di opzioni per il ricollocamento obbligatorio, un programma per il reinsediamento dei profughi e un piano per il rimpatrio degli irregolari. Credo sia opportuno ricordare a tutti noi che il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione. L'articolo 10, terzo comma, prevede infatti che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Questo disegno di legge, già approvato in prima lettura dalla Camera con un'ampia maggioranza, ha un grande valore simbolico, ma non solo: deve costituire anche uno sprone perché l'Unione europea ritrovi quell'elemento costitutivo della solidarietà che era nella mente dei Padri fondatori, ma che sta purtroppo venendo meno nella gestione dell'emergenza dei migranti, un fenomeno epocale che va governato uscendo dalla logica emergenziale e, soprattutto, non lasciando soli i Paesi di primo approdo come l'Italia e la Grecia. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'UNHCR e l'UNICEF, dal mese di settembre del 2015, 340 bambini, in media due al giorno, hanno perso la vita in mare nel tentativo di attraversare con le loro famiglie il Mediterraneo orientale.

dell'associazione UN Women for peace, che è intervenuta martedì 8 marzo a Istanbul a una conferenza sui diritti delle donne, dall'inizio dell'attuale crisi le persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere il nostro continente sarebbero circa 4.000, un numero spaventoso al quale non si può rispondere con l'indifferenza e con l'innalzamento dei muri. Certo, non aiutano l'Europa i vertici come quello del 15 febbraio scorso del Gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria), allargato a Bulgaria e Macedonia e non aiuta la continua minaccia di sospensione del Trattato di Schengen. Nel corso delle celebrazioni del primo anniversario della tragedia di Lampedusa, nel 2014, il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, aveva detto: detto: «Ci siamo riuniti qui a Lampedusa perché siamo consapevoli che nelle nostre politiche di asilo e di migrazione c'è qualcosa che non va. Ma vogliamo correggerle. Credo che non vi sia luogo migliore di Lampedusa per segnare una svolta in queste politiche». In effetti, poi, nel maggio successivo è stata approvata l'Agenda europea sulle migrazioni, che è però rimasta in larga parte inapplicata a causa del risorgere degli egoismi nazionalistici e della crisi generale dell'Unione europea. Prova ne è il difficile vertice con la Turchia di lunedì scorso. Qualche settimana fa, una delegazione della Commissione per i diritti umani del Senato si è recata a Lampedusa, dove ha potuto riscontrare l'impegno degli operatori ma anche le oggettive difficoltà nella realizzazione degli *hotspot*. Auspico che dal dibattito su questo disegno di legge, anche se so che non è semplice, restino fuori le legittime polemiche su come gestire l'immigrazione, perché ha buone ragioni sia chi dice che c'è bisogno dei migranti per contrastare l'invecchiamento della popolazione in Europa e per poter contare su forza lavoro aggiuntiva e su nuovi consumatori, sia chi sostiene che la ragion di Stato impone di non sovrapporre le ragioni di ordine umanitario e le ragioni dell'accoglienza a quelle di chi è convinto che è sbagliato confondere la missione della Chiesa con i compiti degli Stati, fare confusione fra il messaggio evangelico e la politica, fra l'universalismo della Chiesa, che parla a tutti gli uomini, e l'inevitabile particolarismo degli Stati, che rispondono ad un insieme definito di cittadini. Questo disegno di legge non intende dare risposta, né potrebbe farlo, ai tanti e complessi problemi posti dall'arrivo di migliaia di rifugiati, ma più semplicemente e magari efficacemente vuole operare sul piano culturale della coscienza collettiva, nel ricordo di chi fuggiva dalle guerre e dal dolore, di chi sognava un futuro migliore per i propri figli ed è morto durante uno dei tanti viaggi della speranza, nella consapevolezza che una nazione civile deve avere fra le sue ragioni fondanti anche la tutela dei diritti umani. Questo è il senso e la ragione profonda che ispira il disegno di legge n. 1878 «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione», che spero venga approvato dal Senato con la maggioranza più ampia possibile. Presentato alla Camera il 13 novembre 2013, ad un mese dalla tragedia di Lampedusa, primo firmatario l'onorevole Chaouki, Realacci, Iacono e Roberta Agostini, è stato approvato - come ho già ricordato - con una maggioranza molto ampia dall'Assemblea di palazzo Montecitorio lo scorso 15 aprile e trasmesso al Senato il 17 aprile 2015, il giorno prima dell'altra grande tragedia nel Mediterraneo al largo di Lampedusa. Mi permetta, signora Presidente, alcune considerazioni aggiuntive. Le vicende che nel Mediterraneo e lungo le rotte via terra verso l'Europa hanno provocato la morte di migliaia di persone, in fuga da guerre, persecuzioni e miseria, sembravano finalmente aver indotto i Paesi europei a un atteggiamento di maggiore apertura verso il fenomeno migratorio. L'Europa tutta, infatti, è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire con azioni più incisive, garantendo ai Paesi maggiormente coinvolti dai flussi migratori il supporto necessario per creare canali umanitari di ingresso e per contrastare il traffico di esseri umani. C'erano state, nei mesi estivi dello scorso anno, addirittura manifestazioni di solidarietà nei confronti dei rifugiati, in particolare da parte dei cittadini austriaci e tedeschi, che sembravano rappresentare un segno tangibile della nuova sensibilità civile che si stava formando su questi temi, che potrebbe davvero rappresentare un ritorno ai fondamenti identitari dell'Unione europea. Le speranze e le tragedie di quanti, spinti dalla disperazione e dalla miseria, fuggono dai propri Paesi alla ricerca di un'esistenza dignitosa ci parlano anche della nostra storia, degli emigranti italiani che subirono il peso dell'indifferenza e il disprezzo del razzismo. Fare memoria del passato serve per imparare a guardare al futuro con senso critico e a porre rimedio agli errori commessi. Credo che l'Italia il suo compito lo stia svolgendo, l'abbia svolto e lo svolgerà. Non così l'Europa: si sono innalzati muri, prosperano i populismi nazionalistici, prospera la xenofobia, come abbiamo visto nelle elezioni di ieri in Germania. Credo che l'Europa debba ritrovare una spinta solidaristica, innanzitutto rivedendo il regolamento di Dublino, che impone ai soli Paesi di primo approdo l'onere dell'accoglienza dei profughi. Abbiamo assistito, da parte della Commissione europea, a delle vere e proprie contraddizioni: prima si lasciano soli l'Italia e la Grecia e poi le si sanzionano con procedure di infrazione, perché non siamo riusciti a prendere le impronte a tutti i profughi in arrivo

e dalla miseria, ma vuole anche essere una risposta all'indifferenza europea, una risposta che ci riporti ad un sussulto

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è con infinito onore e profondo senso di responsabilità che siamo finalmente riuniti oggi, per approvare un provvedimento da molti mesi in attesa di approvazione da parte di questa Il 3 ottobre 2013 ricevemmo tutti uno schiaffo, dato dalle immagini dei corpi alla deriva di 366 vittime, uomini e donne, morti a pochi metri dalle coste di Lampedusa, migranti che avevano quasi raggiunto la tanto agognata libertà, per la quale avevano investito buona parte dei loro risparmi, messi nelle mani di trafficanti senza scrupoli. Quella tragedia, seppur annunciata perché preceduta e purtroppo seguita da altre vicende di morte e disperazione, ha risvegliato in molte coscienze un senso di responsabilità e vicinanza nei confronti delle tante migliaia di persone, che da anni affrontano la breve traversata che separa le nostre coste dall'Africa, e ha spinto il Parlamento e il Governo a tradurre quello schiaffo in una risposta politica, con la decisione di istituire una giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione. Questa giornata deve servire da monito, come stabilito nel testo di legge che siamo chiamati ad approvare, con il fine di promuovere la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Una giornata nella quale verranno organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini in ordine alla dignità dei migranti, all'importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «L'umanità che mostreremo nell'accogliere i profughi disperati, l'intelligenza con cui affronteremo i fenomeni migratori, la fermezza con cui combatteremo i trafficanti di essere umani saranno il modo con il quale mostreremo al mondo la qualità della vita democratica». Ed è proprio per dimostrare la nostra profonda umanità, la nostra più viva solidarietà, ma anche per dimostrare e per ricordare sia a noi stessi che ai nostri vicini europei che noi Italiani, che in passato siamo stati un popolo di emigranti, non abbiamo dimenticato le nostre origini e oggi vogliamo tendere una mano nei confronti di chi fugge da violenze, guerre e povertà alla ricerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli, Ricordare uomini, donne, bambini, di cui non sappiamo il nome e di cui non conosciamo il passato, non solo ci rende persone migliori, ma ci serve per comprendere che chiudere le porte

accompagna i periodi caratterizzati da forti cicli migratori. Mi auguro che questa giornata possa venir celebrata in un clima di coesione e solidarietà, che non sia solo una passerella autocelebrativa istituzionale, condita dalla solita retorica e demagogia, perché dobbiamo dare ai cittadini, all'Italia e all'Europa risposte concrete, reali e rapide, che sappiano dare una risposta alla richiesta di accoglienza, di solidarietà umana, senza alcuna strumentalizzazione. Il mar Mediterraneo, che è stato per secoli culla di civiltà, oggi è diventato la frontiera che separa i ricchi dai poveri, i fortunati dagli sfortunati, chi ha un futuro da chi non ce l'ha. l'ha. Non voglio e non posso accettare questa suddivisione. Come scrisse più di cinquant'anni fa don Lorenzo Milani, «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io (...) reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri». Bene, io non voglio trovarmi dal lato dei privilegiati, né da quello degli oppressori. Voglio e desidero, per i miei figli e i miei nipoti, un futuro dove la solidarietà, i diritti umani e i valori dell'accoglienza e dell'integrazione siano alla base alla base della convivenza civile. Per questo sono favorevole all'istituzione di questa giornata della memoria, al fine di trasmettere, soprattutto alle più giovani generazioni, i valori dell'integrazione e della fratellanza tra i popoli. Di certo l'Italia, da subito, ha dato dimostrazione di avere a cuore il problema e di volersi impegnare per risolverlo. Lo dimostra il lancio dell'operazione Mare nostrum, voluta dal Governo Letta nelle settimane successive il naufragio, con lo scopo di pattugliare il canale di Sicilia, unendo un obiettivo militare ad uno scopo umanitario ancora più nobile, di voler prestare soccorso ai clandestini evitando il ripetersi di altri tragici incidenti. Che questa giornata sia allora un'occasione anche per ascoltare le testimonianze dei tanti e coraggiosi operatori della Marina militare, della Guardia costiera e delle altre Forze dell'ordine, impegnati da anni nel salvataggio di vite umane, lavorando di notte, al freddo e al vento, instancabilmente, con il solo nobile scopo di aiutare quante più persone possibile, a prescindere dal colore della pelle, dell'origine e della condizione sociale. Ho ancora i brividi nel ricordare le parole e le lacrime di tanti ufficiali intervistati da stampa e televisione in quei tragici giorni, quando tra le lacrime ricordavano gli sforzi fatti, i cadaveri ripescati, i bambini senza più genitori e i genitori senza più figli.

Non ci sono mai state tante persone in fuga da persecuzioni politiche e guerre come oggi e a queste si aggiungono i milioni di migranti economici che premono dall'Africa nera e subsahariana. Molti di loro cercano protezione qui in Europa e solo se riusciremo ad entrare nell'ordine delle idee che questa situazione non cambierà nei prossimi anni, potremo offrire una risposta convincente e risolutiva. Finora, infatti, le risposte messe in campo dall'Europa sono state parziali - lasciatemelo dire - troppo timorose e condizionate dalle situazioni interne ai singoli Stati. Tuttavia, se l'Europa non riesce ad essere all'altezza delle aspettative che tutto il mondo nutre nei suoi confronti, quale diventi lo scopo stesso di stare tutti insieme, se non si è in grado di dare una risposta forte e univoca a un problema globale. Per questo motivo, spero che il Governo voglia perseguire in Europa una politica comune per la gestione non solo dei richiedenti asilo, ma anche dei profughi e degli immigrati economici, basata sul principio di solidarietà e sul nostro valore dell'umanità che noi tutti condividiamo. Non è questa la sede per affrontare il tema dei cambiamenti e delle modifiche che andrebbero introdotte nelle regole europee, tuttavia mi piace pensare che nell'Unione europea che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti i migranti saranno accolti ovunque con eguale dignità umana, attraverso l'introduzione di *standard* minimi validi in tutti i Paesi membri. che i migranti possano essere equamente suddivisi tra tutti i Paesi con un sistema intelligente di quote, che tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro di un'Unione formata da 500 milioni di persone e che quindi può e deve riuscire a gestire un fenomeno migratorio che, pur arrivando al milione di unità all'anno, rappresenterebbe una situazione come quella odierna, in cui il peso della crisi è scaricato tutto sui Paesi di frontiera e su quei pochi, generosi Paesi che, su base volontaria, decidono di offrire accoglienza ai profughi, è destinata a fallire poiché non introduce criteri comprensibili da tutti i cittadini, correndo il rischio di creare tensioni e recriminazioni di vario genere. Chiaramente, nel medio-lungo periodo dobbiamo andare oltre la gestione dell'emergenza, intervenendo sulle cause dell'immigrazione, magari attraverso l'introduzione di accordi di partenariato con i Paesi dell'altra sponda del Mediterraneo da cui transitano i migranti, rafforzando anche ulteriormente il pattugliamento delle coste, il più vicino possibile ai porti dei Paesi nordafricani dai quali salpano i barconi, ma sempre agendo come Unione europea e non come Italia, Grecia o Spagna. Per riuscire a creare una politica di accoglienza a tutto campo dobbiamo incoraggiare delle iniziative politiche che combattano le ragioni alla base dell'emigrazione dai Paesi del Medio Oriente e dell'Africa. La stabilizzazione della situazione di Stati che si stanno sfaldando, la limitazione di violenza e guerre civili devono procedere di pari passo con precisi sforzi che supportino lo sviluppo economico e la creazione e la creazione di reali prospettive economiche e sociali, in special modo per i tanti giovani cittadini di quelle nazioni, se non vogliamo che a decine di milioni, nei prossimi anni, Tutti gli sforzi delle comunità di Stati, innanzitutto dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, devono avere questo scopo. Spero quindi che l'Europa, chiamata ad assumersi le proprie responsabilità, decida di non lasciare soli i Paesi di frontiera come l'Italia e la Grecia, e possa garantire ai Paesi più coinvolti dai fenomeni migratori, principalmente per motivi geografici, tutto il supporto necessario al fine di gestire con maggiore efficacia i numerosi sbarchi, modificando anzitutto la norma sul diritto di asilo contenuta nel Regolamento di Dublino del 2008, con l'introduzione di quote proporzionali che superino il vincolo del primo Paese di ingresso nell'Unione, oggi troppo penalizzante per i Paesi mediterranei. I cittadini europei si sono già dimostrati sensibili a queste tematiche, con manifestazioni di solidarietà, segnali concreti di una nuova sensibilità civile che si sta formando su

muri che si alzano e frontiere che si chiudono. Spetta allora ai Governi - e mi auguro che il Governo italiano possa farsene portavoce - creare un'Europa più solidale nei confronti dei migranti, che possa dare risposte concrete, reali e rapide alla richiesta di accoglienza e di solidarietà umana che giunge dai suoi confini. Voglio concludere, signora Presidente, ribadendo il mio sostegno all'introduzione di questa giornata della memoria, ricordando una frase pronunciata da un giovane rifugiato che disse: «Non sono pericoloso, sono in pericolo». Ebbene non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte quando riceviamo queste richieste di aiuto, dobbiamo invece offrire il nostro sostegno e la nostra solidarietà, tenendo a mente le parole di Papa Francesco quando denuncia la globalizzazione dell'indifferenza quale male della nostra epoca e della nostra società, perché questo è ciò che vorremmo ricevere, se un giorno ci trovassimo noi nella stessa situazione. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge di cui stiamo discutendo riconosce il 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, con lo scopo di sensibilizzare e formare l'opinione pubblica e le giovani generazioni alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e al valore della vita. Quella data - il 3 ottobre - è impressa nei nostri cuori, quelle immagini ci sembrarono insopportabili e speravamo di non doverle più vedere ma così non è stato e, forse, ci siamo anche un po' rassegnati a tutto questo e solo di tanto in tanto l'immagine di un piccolo tra le braccia di un soccorritore che arriva - ahimè - troppo tardi ci costringe a riflettere. È di qualche giorno fa la nascita di un piccolo venuto alla luce in mezzo al fango: tutti abbiamo davanti agli occhi quell'immagine. Ho pensato, nei giorni scorsi, che, almeno, Gesù bambino, quando è nato, aveva il bue e l'asinello a riscaldarlo, mentre quel bambino non aveva neanche questo. Integrazione, accoglienza e inclusività: sono questi i pilastri concettuali su cui si fondano gli eventi che saranno organizzati nel giorno della memoria. Non dunque, colleghi, mero ricordo di una tragedia che inevitabilmente ha scosso le anime di tutti i cittadini e le cittadine, che hanno vissuto con ansia e apprensione quelle drammatiche ore in cui le notizie riportavano un numero di morti sempre crescente. Vorrei rimarcare il significato più profondo che rappresenta l'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione: promuovere l'educazione dei nostri ragazzi nelle scuole e dei cittadini e delle cittadine nei luoghi in cui vivono. È questo un investimento culturale per il futuro del nostro Paese, che potrà, spero, contagiare gli altri Paesi europei

Ma torniamo a noi. Ogni singolo membro della società civile è portatore di valori e consuetudini che si riflettono sulla collettività e ogni azione positiva rivolta all'inclusione deve essere scientemente accolta. Questo è un modo concreto di supportare quegli intenti di cui l'Italia si sta facendo portavoce presso le istituzioni sovranazionali e aiuta a compiere quel passettino in avanti, cui ha fatto riferimento il nostro *Premier* all'ultimo Consiglio europeo, che guarda alla sostanziale rivisitazione delle politiche comunitarie in tema di accoglienza e solidarietà. Ridare alle istituzioni europee quel senso di umanità, quel cuore sempre più spesso sostituito dal calcolo dei vincoli finanziari, è una priorità per non alimentare ulteriormente le ragioni di chi disconosce i benefici di una comunità che necessita urgentemente di una reale ed inderogabile integrazione culturale. Ogni azione, compresa l'istituzione di una Giornata di ricordo per le vittime di Lampedusa nel 2013, deve servire a far riflettere sui numeri dietro cui si celano le storie personali e familiari di uomini, donne e bambini.

Nel 2015 sono stati oltre 3.500, di cui 800 bambini: cifre da rabbrividire. Ma le cifre non ci raccontano i volti, gli sguardi, gli occhi di quelle persone che cercano una vita più dignitosa. Morti nel Mediterraneo: un mare che è stato culla di scambi culturali nei secoli scorsi e che, nella visione profetica di La Pira, doveva rappresentare un ponte, quel "lago di Tiberiade". E invece questo mare si è tinto di rosso, delle tante vite perse di uomini e donne che cercavano solo una vita più dignitosa. Ma voglio rinforzare il concetto di poc'anzi: non possiamo permettere, come Paese, che l'Europa scarichi sulla buona volontà e sul senso di accoglienza di piccole comunità come Lampedusa, Augusta, Pozzallo - per ricordare soltanto le più note - l'onere di una responsabilità politica molto grande. In quelle comunità non si parla né di numeri, né di paura, perché non c'è tempo. Esse sono il simbolo di una generosità e di una solidarietà che davvero fanno da ponte fra culture diverse, offrendo, a chi li cerca disperatamente, aiuto e sostegno. L'idea di dare il premio Nobel per la pace a Lampedusa è un'iniziativa assolutamente lodevole, perché protesa all'idea di un'Europa il cui cuore pulsante batta in mezzo alle persone. Tale idea rappresenta una spinta concreta a favore della nostra posizione in sede europea, per una rivisitazione del Regolamento di Dublino, per l'introduzione di una gestione comune dell'asilo, per convincere dei benefici e non delle minacce e delle paure della libera circolazione. Rappresenta, cioè, una modalità per far crescere nella consapevolezza della necessità di accoglienza quelle comunità le cui risposte sono racchiuse nell'arroccamento e nella chiusura. Non lasciamo che prevalgano l'austerità severa e le finalità utilitaristiche nella visione di un'Europa che rischia fortemente di piegarsi su se stessa, di spegnersi, e che lascia nei sentimenti degli italiani quei numeri inquietanti per cui solo il 13 per cento della società sarebbe favorevole alla libera circolazione nell'area Schengen. L'ammonimento lanciato da Marco Impagliazzo nei giorni scorsi in un editoriale su «Avvenire» la settimana scorsa, per evitare che una nuova cortina di ferro cali sull'Europa, ci deve far riflettere a lungo su come la storia possa, mutate le circostanze, obnubilare le menti e far perdere di vista quei poli culturali cui abbiamo deciso di aderire con convinzione e che sono alla base del nostro sistema democratico, fondato su temi quali l'inclusività, la solidarietà, la speranza, l'accoglienza, l'uguaglianza, il diritto alla vita e alla salute. Governare i flussi migratori secondo un'ottica che privilegi queste tematiche è una sfida, certamente complessa, che riguarderà anche i prossimi anni, anni, alla quale ad ogni modo bisognerà rispondere. Spero in questo senso che si acceleri la creazione di condizioni migliori per dare inizio ad un reale processo di inclusione culturale e umanitaria, scevro da derive o tentazioni populiste. I recenti numeri del fenomeno migratorio ci riportano, dati alla mano, alla realtà di dover affrontare un fatto imponente: per Frontex sono stati 170.000 gli arrivi di migranti in Italia nel 2015; per l'ONU 9.000 solo in questi primi due mesi del 2016. La proposta delle istituzioni europee di creare una guardia costiera e di frontiera europea, che è all'attenzione del Parlamento, e la scelta della Commissione per un percorso di ripristino di Schengen indicano la direzione di attuazione dei pilastri dell'Agenda europea sulla migrazione del 2015, soprattutto sull'idea della gestione comune di flussi di migranti. Se tutto questo può essere utile per evitare al massimo il possibile ripetersi di episodi come quello di Lampedusa del 2013, ben intervenga l'Europa in aiuto degli Stati nazionali e di quelle popolazioni che, per ragioni geografiche, si trovano in prima linea. Tali possibili argini, però, non si sleghino da esigenze umanitarie, restando soltanto soluzioni di facciata. Senza la convinzione che lo sviluppo del sistema di accoglienza deve essere integrato e la gestione delle responsabilità condivisa, difficilmente si potranno trovare soluzioni soddisfacenti per la gestione dei flussi migratori. In quest'ottica va certamente accolta con favore la risoluzione, approvata nei giorni scorsi dal Parlamento europeo, che sostiene che la violenza di genere dovrebbe essere un valido motivo per richiedere l'asilo nell'Unione: proteggere i bambini e le donne vittime di violenza o di tratta di esseri umani, è uno dei compiti più importanti che un sistema comune deve assicurare. Papa Francesco, il 17 gennaio scorso, giorno del Giubileo dei migranti, ha ricordato come ognuno porti con sé «una storia, una cultura, dei valori preziosi; e, spesso purtroppo anche esperienze di miseria, di oppressione, di paura». Il Santo Padre ci ricorda come attualmente, più che in tempi passati, «il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, impedisce che ci si abitui alla sofferenza dell'altro e indica vie di risposta» che possono declinarsi «nelle opere di misericordia spirituale e culturale». Ha aggiunto che è importante, quindi, «guardare ai migranti non soltanto in base alla loro condizione di regolarità o irregolarità ma, soprattutto, come persone che, tutelate nella loro dignità, possono contribuire al benessere e al progresso di tutti», proprio per non ridurre le migrazioni a fenomeni meramente economici, normativi, politici. «Questi aspetti sono complementari alla difesa e alla promozione della persona umana, alla cultura dell'incontro dei popoli e dell'unità». Solidarietà e comprensione siano, allora, i valori cardine su cui ripartire per affrontare l'intera questione dell'accoglienza, istituzioni e società civile.

Oltre le visioni utopistiche, in quanto al di là delle soluzioni prospettate è difficile che si riduca la portata dei flussi migratori sui Paesi di frontiera membri dell'Unione, si può ripartire da progetti concreti che evitino al massimo che tragedie come quelle del 3 ottobre 2013 possano accadere di nuovo.

che detta ricorrenza possa apparire una strumentalizzazione dell'immensa tragedia di Lampedusa al fine di mettere in campo l'ennesima operazione di facciata. Non punto il dito contro nessuno. L'atteggiamento celebrativo spesso nasconde pratiche farisaiche, un agire consapevolmente ipocrita da parte del ceto politico di fronte a responsabilità collettive,

Grazie queste immani tragedie e contrastare efficacemente la clandestinità, l'illegalità e i trafficanti di esseri umani. L'istituzione della Giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione, a nostro avviso, se non accompagnata da un concreto cambio di passo nelle azioni di contrasto alle organizzazioni criminali al traffico di profughi, può rappresentare solo una pelosa elargizione di compassione che nasconde l'incapacità del Governo di incidere sulle cause del fenomeno migratorio; e tanto meno responsabilizza l'Europa nelle fasi iniziali dei processi migratori, adottando misure che sarebbero necessarie, quali l'accoglienza *pro quota* dei migranti da parte degli Stati membri. Il cambio di passo prevede l'assunzione di responsabilità dell'Europa a 28, affinché i popoli europei riconoscano, solidalmente consapevoli, che ci si salva insieme e che insieme ci si occupa di un fenomeno dai tratti biblici epocali. L'esodo può essere frenato alla radice, a monte: nei luoghi in cui origina il disagio, opponendo politiche che prevedano investimenti comunitari in risorse umane, professionali, tecnologiche, finanziarie, per garantire migliori condizioni di vita, prospettive di sviluppo, creazione di nuovi mercati e nuove professionalità, in grado di contribuire al progresso di quei popoli, di quegli Stati, oggi drammaticamente sotto sotto la soglia della povertà. Certamente non possiamo non condividere il concetto di memoria quando è la memoria nazionale della nostra storia, dei nostri martiri, del ricordo di un passato che serve per imparare a guardare al futuro con senso critico, sensibilizzare, e porre rimedio agli errori commessi. In questo caso specifico, però, la memoria sembra non avere nulla a che fare con questo tipo di suggestione; piuttosto, sembrerebbe avere il sapore dell'ennesimo specchietto per le allodole predisposto dalle forze politiche presenti in Parlamento, troppo spesso diligenti ad organizzare cerimonie e iniziative con buoni propositi che nascondono un'oscura opera di proselitismo e di pura propaganda politica. Senza contare che forse troppo spesso ci appelliamo alla sensibilità degli italiani, dimenticandoci, più o meno intenzionalmente, di sollecitare la sensibilità per gli oscuri oscuri eroi della nostra recente storia e per gli eroi di oggi, che ogni giorno sono vittime dell'incuria di uno Stato e di una politica sempre meno attenta e sensibile alle tragedie dei propri cittadini. Tutti coloro, insomma, che non sono commemorati in alcun modo, proprio come le nostre vittime dell''immigrazione, coloro che negli anni Sessanta, numerosi, dal Sud e dalle Isole emigrarono verso il Settentrione. Oppure quella decina di milioni di emigrati italiani che, dagli inizi del Novecento, sono espatriati, soprattutto dal nostro Mezzogiorno o dalle sacche indigenti del Nord e del Centro, verso gli Stati Uniti e, nel secondo dopoguerra, verso la Germania e gli Stati ricchi di materie prime come Francia, Benelux e Svizzera. Anche qui, migliaia di morti, condizioni di lavoro inumane, baratto di Stato tra forza lavoro per le attività estrattive estrattive e carbone per alimentare l'industria pesante, drammi famigliari, distacco penoso, depauperamento drammatico del tessuto sociale, affettivo, economico e produttivo dei nostri Paesi e delle nostre campagne.

Sollecitiamo altresì diligentemente, dai banchi dei due rami del Parlamento, l'istituzione presso l'ONU di identica iniziativa politica, con il pensiero rivolto all'immane dolore dell'umanità che perde migliaia di piccoli, adolescenti, bambine e bambini, inghiottiti dal mar Mediterraneo nelle difficili traversate. È divenuta virale la foto di un piccolo naufrago che giace su una remota spiaggia in Turchia: il corpicino di Aylan, raccolto

Vorrei aggiungere qualche mia osservazione, richiamandomi all'alto valore di questo disegno di legge, che istituisce la Giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione,

una comunità accogliente e che si sta pesantemente dividendo su valori che pensavamo fossero le pietre angolari e costitutive del sogno europeo. vogliamo ancora tenere forte e fermo questo sogno. Vorrei proseguire con una frase del presidente Donald Tusk, il quale mi ha francamente molto colpita e anche sorpresa quando ha annunciato

fondatori di riconoscersi per origini comuni cittadini di un unico continente geografico e culturale? Sembra quasi incredibile il punto di arrivo. Oggi vediamo avanzare spinte nuove, ma con una velocità e con un modo quasi uniformemente accelerato: mi riferisco a spinte nazionalistiche, rigurgiti xenofobi e pulsioni incivili

Verso persone che vanno alla ricerca di un varco verso la speranza. Certi video hanno lasciato in questi giorni la società civile sconcertata. civile sconcertata. Perché l'Europa con le sue istituzioni democratiche mette all'angolo principi solidaristici? Perché non procede con una politica seria di *relocation*, richiamata più volte dal relatore? Perché non agisce

L'Italia ha fatto e sta ancora facendo la sua parte in prima linea per un'efficace politica di accoglienza per identificare i migranti e gestirne il flusso, per accelerare le procedure per il ricollocamento, a prescindere da restrizioni, senza discriminazione, sulla base della nazionalità. L'Italia si impegna in una politica non adeguatamente riconosciuta dall'Europa. Abbiamo

migranti. Questi non devono però trasformarsi in una struttura afflittiva, quasi semicarceraria, dove queste persone

Ecco, dunque, l'importanza di testimoniare con questo provvedimento la nostra attenzione quotidiana nei confronti di popolazioni in sofferenza che vedono nell'Europa il sogno di un futuro possibile e non la dannazione. Per tutti coloro che nei viaggi della speranza hanno perso la vita in mare (20.000 persone solo negli ultimi anni), la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione è un evento e una celebrazione dovuta e commossa. È una giornata che,

per una risposta - bene ha detto il relatore Mazzoni - all'indifferenza. Affinché tutti gli studenti, dal mondo dell'infanzia a quello dell'adolescenza, comprendano il valore dell'uomo e riflettano,

pensino e si immedesimino nel dramma e nella sofferenza che si nasconde dietro alla parola. La fuga dalla guerra e dalla morte per cercare la vita non è solo il frutto di un desidero legittimo, ma è espressione di un diritto inviolabile. Ma questa sfera dei diritti sembra davvero sfuggire a più di qualcuno.

Vorrei invitarvi, colleghe e colleghi, signora Presidente, a guardare un po' indietro, per capire perché lo ritengo un dovere morale e politico. Voglio invitarvi a guardare alla nostra storia e non voglio utilizzare parole mie, ma mi permetterò di leggere alcuni Voglio leggervi alcuni pezzi di un articolo pubblicato su «la Repubblica» il 28 agosto 2009 dalla giornalista Giulia Vola, durante un suo viaggio nel mondo ha incontrato dei nostri emigrati: «Buenos Aires. "Buttarono nell'Oceano donne, un bambino e molti vecchi, in tutto quasi venti persone. Così raccontava mio padre". Maria Dominga Ferrero vive in provincia di Cordoba, in Argentina, nella casa che suo padre comprò quando, nel 1888, arrivò alla "Merica"» - si chiamava "Merica" allora, nel linguaggio dei nostri migranti - «a bordo del Matteo Bruzzo. Maria parla un po' in piemontese e un po' in castigliano, mentre gira la minestra di verdure che bolle sul fuoco. "La solfa era la stessa. La differenza era che se sopportavi il male potevi fare *suerte*, fortuna. Non come capita agli immigrati che oggi vanno in Italia"». Lo dice la figlia di un nostro primo emigrante. prosegue: «Felicia Cardano è molto anziana, ma ricorda bene i racconti di famiglia: "Mio padre arrivò a Buenos Aires nel 1889 a bordo del Frisca. Durante il viaggio morirono il suo migliore amico e altre trenta persone. Lo misero all'Hotel un enorme baraccone di legno, dove si stava stipati come sardine insieme ai pidocchi e alla puzza. Si poteva rimanere al massimo cinque giorni, il tempo di trovare un lavoro in città

ha una forma strana, sembra un gasometro munito di finestre (...). L'acre odore dell'acido fenico non riesce a vincere il tanfo nauseante che viene dal pavimento viscido e sporco».

Noi, vittime di allora, fuggivamo dalla Grande Guerra. Racconta Margherita Lombardi, nipote di Clelia scappata da Alessandria: "Mia zia perse un figlio in battaglia nel 1916 e un altro nel viaggio sull'Oceano. Si salvò solo lei"». Come dicevano con terrore le madri: «"Meglio un figlio lontano ma vivo che vicino ma sotto terra, disse mia nonna a mio padre Fernando"». Altre testimonianze: «"Ci imbarcammo sulla Filippa senza documenti e senza un soldo il giorno dopo che Miguel tornò dal campo di concentramento in Germania"». Altra testimonianza: «"Mio padre scappò da Fossano e dalla guerra che gli aveva ucciso un fratello - racconta Antonio Caballero - , aveva 17 anni e fin dal primo giorno cominciò a dimenticare l'Italia. Non ho mai parlato con i miei parenti rimasti a casa. Non ho mai imparato l'italiano perché nessuno me l'ha mai insegnato. Nessuno di noi ha fatto fortuna, semplicemente siamo sopravvissuti"». I poeti popolari del Meridione italiano hanno parlato di questa storia e Vigo, nel 1970, chiamò il momento della partenza dell'emigrante «spartenza», ovvero separazione, per indicare un distacco violento e doloroso. Durante il viaggio, però, gli emigranti spesso non avevano tanto tempo per la meraviglia, la noia o la nostalgia: c'erano il mal di mare, l'indifferenza e gli abusi dell'equipaggio, la paura dei naufragi e delle malattie contagiose e la possibilità di essere sbarcati in un Paese diverso da quello previsto. Gli italiani erano privi di un'efficace protezione da parte della legge e le speculazioni delle compagnie di navigazione potevano trasformare il viaggio transoceanico in un'esperienza altamente rischiosa. II trasporto di emigranti fu un grosso affare per la marina mercantile italiana. nel 1894, Edmondo De Amicis viaggiò da Genova all'Argentina, a bordo del piroscafo Nord America, insieme a 1.600 emigranti italiani. Pubblicato nel 1889, il romanzo «Sull'oceano», che racconta i ventidue giorni di quel viaggio, ottenne uno straordinario successo e divenne un modello obbligato per coloro che si accingevano a scrivere della traversata transoceanica. Sia nelle situazioni che nella scelta lessicale, lo scrittore ligure utilizza l'immagine classica dell'inferno dantesco per descrivere la condizione di estrema sofferenza dei passeggeri di terza classe. Questo modello letterario è stato spesso adottato dagli stessi emigranti, in riferimento alla propria esperienza: «Se Dante avesse conosciuto ciò che erano le terze classi dei transatlantici nel 1885, per certo ne avrebbe descritta una e l'avrebbe allogata nell'inferno e vi avrebbe inchiodato i peccatori de' più neri peccati». Il viaggio verso il nuovo mondo durava dalle due alle quattro settimane, in base alle condizioni del mare e al carico. Durante questo periodo, l'affollamento e la sporcizia dei dormitori diventavano tali da spingere l'igienista Vittorio Cantù a scrivere che «l'impressione di disgustosa ripugnanza che si riceve scendendo in una stiva dove hanno dormito gli emigranti è tale che, provata una volta sola, non si dimentica più».

«Me la strapparono dalle braccia, la fasciarono stretta stretta da capo a piedi e le legarono una grossa pietra al collo; di notte, alle due di notte, con quelle onde così nere, la calarono giù in mare. Io urlavo, urlavo non volevo staccarmi da lei, volevo annegare con la mia piccola (...). Non volevo lasciarla sola, povera bambina, invece mi tennero indietro mentre la buttavano giù.

pensavo che non utilizzando parole mie, avrei annoiato di meno l'Assemblea, ma vedo che non è così. Per quanto tremende potessero essere le condizioni di viaggio, molto spesso, però, la principale preoccupazione dei passeggeri era che la nave sarebbe affondata. Gli emigranti italiani furono coinvolti in decine di naufragi,

è così cambiato? La situazione delle persone, dei bambini, delle donne e degli uomini

in quegli anni la nostra invasione della Svizzera fece nascere i primi movimenti politici xenofobi. Chi ha i capelli bianchi come me ricorderà un nome difficilmente pronunciabile in italiano: Schwarzenbach. Schwarzenbach. Egli era un deputato, un uomo politico che fece votare il popolo svizzero sulle prime iniziative non antistraniere, ma antitaliane

Eppure oggi in quel Paese, che era a rischio di invasione di italiani, la nostra seconda generazione fa parte integrante della classe dirigente: oggi i

Io credo che non ci sia molta differenza tra mio padre, che lasciò l'Abruzzo facendo i debiti per pagare il biglietto del treno (perché non aveva neanche quelle risorse) e andò in Svizzera per far stare meglio mia

colpito quella città erano tutti emigranti stranieri: di fatto erano francesi e belgi, ovvero cittadini europei nati in Europa; erano figli di emigrati. Come è possibile allora una cosa del genere? Perché vogliamo rimuovere questa realtà senza riflettere?

La parola «integrazione» meriterebbe un dibattito in quest'Aula e nel mondo politico italiano, per quello che ci riguarda, e lo meriterebbe anche sul piano europeo, come ricordava prima il collega Liuzzi. che non c'è nessun buonismo nelle mie parole perché sarebbe troppo comodo e troppo facile e io credo che il vero nemico dell'integrazione, il vero nemico della possibilità di affrontare con serietà questi temi sia proprio il buonismo. Nella parola «integrazione» il buonismo non esiste. «Integrazione» è una parola complicata, è una parola nella quale si può mettere tutto e il contrario di tutto, ma dovremmo metterci d'accordo, un giorno, su cosa dovrebbe contenere. Dobbiamo guardare il resto del mondo e il resto dell'Europa per quello che hanno fatto, per le cose buone e le cose cattive che abbiamo fatto in Europa. esempio la Francia, per anni, ha sostenuto che l'integrazione non era una strada percorribile, ma che la strada giusta era l'*assimilation*, l'*assimilation*, che vuol dire che se io arrivo in Francia devo assimilarmi ai francesi. Gli inglesi hanno sostenuto un'altra teoria, non so neanche bene come definirla: la multietnicità, salvo accorgersi che nelle periferie inglesi scoppiano degli scontri perché quando una comunità vive richiusa su se stesse non è integrata. La parola «integrazione» non si può lasciare ai sociologi e agli specialisti. La parola «integrazione» riguarda la società, l'insieme delle politiche,

che rispettino la nostra storia che è ricca di esperienze di emigrazione? Io credo che questo dovremmo fare e se lo facciamo con serietà allora alla parola «integrazione» si può tentare di dare un senso.

abbiamo fatto in un piccolo Paese non europeo, la Svizzera, dove sono invecchiato. Qualche anno fa, nel 2002, le associazioni degli stranieri residenti in Svizzera

problema è proprio quello: integrazione vuol dire che io, straniero, non arrivo in un deserto da conquistare, ma in una società che ha i suoi valori

che hanno un destino comune: costruire una società migliore di quella in cui viviamo oggi. La parola «integrazione» ci richiama alle nostre politiche, alla *Realpolitik*. Io, che non sono della famiglia politica della cancelliera tedesca Merkel, non posso tuttavia non esprimere grande rispetto per la sua reazione al voto di domenica in Germania.

ci richiama anche a questo, ad una vera politica di cooperazione allo sviluppo. E la politica di cooperazione allo sviluppo non può essere determinata

Signora Presidente, ciò che avvenne il 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa fu indubbiamente una gravissima tragedia: morirono

le vicende drammatiche, i naufragi che avvengono ancora in questi giorni? È evidente a tutti che il provvedimento non inciderà minimamente rispetto a questi fatti tragici. la domanda a cui dobbiamo rispondere è a cosa esso serve. Se non ha alcun effetto tangibile, immediato per evitare siffatte tragedie, qual è il motivo per il quale

cerimonie finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza.

È evidente che quella giornata sarà inevitabilmente dedicata alla propaganda sulle politiche dell'immigrazione della sinistra, del Partito Democratico e di questo Governo. Non avrà alcun effetto concreto nel salvare vite umane, ma avrà esclusivamente l'obiettivo di educare i giovani ad una visione del tema dell'immigrazione così come impostata da una parte politica. Noi riteniamo evidentemente che l'ipocrisia che sta alla base del provvedimento sia assolutamente inaccettabile, che serva esclusivamente ad una parte politica per affermare le proprie visioni rispetto ad un tema così grave che riguarda la nostra società, il nostro Paese, l'Europa intera negli ultimi anni. Dovremmo poi chiederci: ma la politica che è stata attuata da questo Governo, quella dell'accoglienza e dei viaggi della speranza (delle false speranze),

di migliaia di persone ad attraversare il mare e ad aver determinato la morte di tutti i migranti? A tale quesito non si risponderà in quella giornata, perché in essa ci sarà una visione unica ed esclusiva, la vostra, quella della vostra maggioranza, quella secondo la quale l'unico motivo per cui sono avvenute le morti è perché la nostra società non è abbastanza sensibile al tema dell'accoglienza e dell'integrazione. Ma non è così. così. È assolutamente falso. Noi siamo contrari che nelle scuole si voglia affermare il pensiero unico portato avanti dalla vostra visione della società, della società, condito da ipocrisia, falsità e falso buonismo, che non rappresenta ciò che dovrebbe essere fatto dal nostro Paese per evitare effetti così tragici. Negare la drammaticità della presenza di vittime e morti alla propaganda e al sostegno di una specifica politica sull'immigrazione è un atto assolutamente fuorviante e meschino. Sfruttare i buoni sentimenti dell'opinione pubblica per fare propaganda è insopportabile e rappresenta - ad avviso mio e della Lega Nord - una forma di cinismo che forse è peggiore di quella degli indifferenti rispetto a simili tragedie umane. Questo provvedimento non è utile a nessuno: non è utile ai migranti, al nostro Paese e ai nostri cittadini. È utile, forse, esclusivamente a una parte politica che avrà la possibilità, in una giornata dell'anno, di affermare nelle scuole e nelle cerimonie che vorrà realizzare su tutto il territorio nazionale la propria esclusiva visione sul tema dell'immigrazione. Quella sarà la giornata della propaganda del Partito Democratico. Per questi motivi la Lega Nord non vuole accodarsi ai dibattiti che si sono svolti e mescolare temi molto diversi, quale la migrazione

dopo la Prima guerra mondiale con le migrazioni di oggi: sono due fenomeni totalmente diversi, che non vanno assolutamente assimilati e non possono essere paragonati. essi si sta cercando solo di creare nello stato d'animo delle persone che hanno vissuto quei fenomeni o ne hanno ricordo la percezione che dobbiamo essere solidali e

di due temi totalmente diversi, che vanno tenuti saldamente distinti. La Lega Nord non condivide questo dibattito; non condivide il fatto che si tenga impegnato il Parlamento su siffatti temi; non capisce perché la Giornata delle vittime dell'immigrazione abbia più dignità della Giornata delle vittime della crisi economica (che sono purtroppo tante) o del terrorismo. È evidente quindi che alla base di questo provvedimento c'è solo ed esclusivamente una cinica propaganda. Anche se fossimo l'unica forza politica contraria al provvedimento, noi vogliamo affermare la nostra contrarietà e diciamo no alle meschinità e all'ipocrisia che stiamo ascoltando in questo inutile dibattito parlamentare. *(Applausi

desidero intervenire offrendo ai colleghi senatori, alla Presidenza e ai rappresentanti del Governo, una riflessione diversa, una riflessione, cioè, che non cada in quel facile piano scivoloso, in quello *slippery slope*, alla luce del quale, evidentemente, una qualsiasi tematica che venga trattata, per quanto nobile sia e per quanto ispirata da più alti valori, possa decadere, possa miseramente scivolare, in una dimensione squisitamente politica, se non di ordine partitico, Per questo motivo, io ritengo che l'intuizione di poter istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime della immigrazione

che si possa cadere in quell'oblio che è una caratteristica propria delle dimensioni umane e che, evidentemente, dà luogo anche a una sorta di psicologica rimozione

di una Giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione ha un significato simbolico. Vorrei ancora una volta richiamare l'etimologia della parola simbolo che - come ci hanno insegnato i greci

Ha un suo simbolismo anche, non a caso, signora Presidente, che la data venga ad essere definita nel 3 di ottobre, in ricordo di centinaia di migranti morti a largo di Lampedusa. Voler ricordare quelle centinaia significa non nascondere le migliaia e migliaia di morti verificatesi nel Mediterraneo,

cercano di raggiungere delle terre che possano assicurare loro libertà, una civiltà, una democrazia, una sufficiente possibilità di vivere. Ed è abbastanza significativo non solo descrivere, ma vivere quelle immagini che vengono non solo dalla zona dei Balcani. Se andassimo a tuffarci anche in altri mari e in alcune zone del nostro grande Mediterraneo,

Così non è e così non deve essere per un motivo e un dato squisitamente oggettivi, che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Noi stiamo assistendo a un fenomeno storico, a una migrazione ineluttabile che segnerà il passaggio, la diversità e il cambiamento il cambiamento del nostro vivere sociale. E se poi questo cambiamento deve caratterizzarsi per centinaia e migliaia di morti, la nostra civiltà, la nostra democrazia e la nostra etica sociale ci impongono, non solo di ricordarle ma, evidentemente, di mettere in essere tutte quelle azioni tutte quelle azioni che diano la possibilità che questo non accada mai più. Qualcuno - è vero - in quest'Aula mi potrebbe dire che si tratta di un'utopia, di un sogno, di una facile speranza.

fondativa dell'esistenza umana. Tengo particolarmente a sottolineare e a porre alla vostra attenzione il fatto che l'uomo è costitutivamente relazionale: è nella relazione dell'altro, nell'incontro con un io o con un tu che si realizza quella prima persona plurale che rappresenta la civiltà,

nobile (vale a dire quella della reciprocità) esiste non più la declinazione di essere con un altro, ma l'altra declinazione della vita, cioè di essere per un altro. E nella dimensione di essere per un altro, io non sarò più - come direbbe Leibniz

*dominus* assoluto, imperatore intangibile e inavvicinabile, ma inevitabilmente sarò solo. Nella dimensione della solitudine, nell'assenza della reciprocità e non della interrelazione, nell'assenza di essere per l'altro, non c'è civiltà, non c'è rapporto sociale, non c'è alterità, non c'è comunione sociale, non c'è comunità. E la comunità non si può costituire tra persone che si sentono uguali tra loro: la comunità si costruisce, si fonda e si elabora in ragione di quella diversità o, più correttamente, di quella alterità che rappresenta la dimensione di essere altro e oltre. Nella dimensione di essere altro e oltre

un filosofo nell'ambito della filosofia del diritto - noi viviamo in una società dove ci consideriamo tutti stranieri morali. Nella dimensione dell'estraneità morale vige una sola legge: chi è più forte rispetto all'altro. Nella dimensione, invece, della costruzione e del superamento dello straniero morale in amico morale, io e te cammineremo insieme. Allora, non saremo più

tante porte. Facciamo l'opposto di quello che diceva Leibniz: io non sarò più una monade, un imperatore incontrastato; non avrò bisogno né di mura, né di fila spinato; io avrò bisogno dell'altro, perché è proprio nell'altro che costruisco la mia identità.

tra soggetti si basa sulla reciprocità. Non si può essere solidali con se stessi, perché peccheremo di quella egoità e di quell'egoismo

politica - è etica della convivenza, del convivere, vale a dire etica dello stare con l'altro e del costruire insieme il percorso del rispetto della dignità umana.

di esigenza storica ed etica di opportunità e utilitarismo, riconoscere o disconoscere ad un altro essere umano la sua dignità. Ma è altra quella che caratterizza ogni essere umano e viene definita dignità intrinseca. Quest'ultima è patrimonio di ognuno e di tutti. Essendo, quindi, una dignità intrinseca, non può non essere riconosciuta; non può non essere fatta valere, non attribuita o evidenziata, ma riconosciuta a tutti i soggetti che pur presentano caratteristiche esterne diverse e che vengono da realtà sociali dovere. La dignità non è un qualcosa che io, Stato più forte, posso o meno riconoscere a un essere umano che viene che viene dalla Siria o dall'Africa subsahariana. Egli è già di per sé portatore di dignità intrinseca, perché la dignità è scritta nella vera e propria

come una posizione *ex* cattedra di chi vuole che gli altri si integrano in ragione di un riconoscimento di distacco come se fossero quegli stranieri cui si concede la possibilità di potersi integrare. Ci si può, però, integrare attraverso una norma di legge; ci si può integrare attraverso un decreto, un dispositivo, un provvedimento; ma ciò è parziale, perché contingente all'aspetto legislativo. La vera integrazione ha bisogno di un valore etico di fondo, quella che viene chiamata interazione, perché solo e soltanto attraverso la interazione noi possiamo - è un passaggio a me caro integrarci reciprocamente. La integrazione non è un *plus* da parte di qualcuno nei confronti di chi, altro, rappresenti un *minus.* Rappresenta in realtà, nella complementarietà propria che caratterizza la natura umana, la dimensione della reciprocità che, attraverso la

Significano saper riconoscere tutti coloro che hanno realmente un bisogno di aiuto. E il bisogno di aiuto nasce da sofferenze e disagi. Non è facile per il vero vorrei ricordarlo a quest'Aula, che su alcuni temi a volte, per ragioni partitiche o correntizie, è un po' distratta - incontrare un quindicenne

affastellate l'una all'altra, senza avere nemmeno la possibilità di uno spazio vitale e di potersi sedere. Se mi dite che, nei confronti di queste di queste persone, di questa umanità, non deve esserci la parola «accoglienza» e non deve esserci il ricordo, delle due l'una: o noi siamo fuori tempo o qualcun altro è fuori tempo in maniera molto, ma molto grave. Credo questo sia uno degli altri aspetti che rappresenta il fondamento di quello che viene definito a me sembra in maniera forte - l'indifferentismo morale. Non è buonismo questo. L'indifferentismo morale significa essenzialmente ritenere che tutto poi passi, che tutto non abbia un valore. Il problema e la criticità di determinate tematiche appartengono solo all'altro, a quel vicino di casa, casa, forse, che avrà un colore di pelle completamente diverso dal nostro, o a quella comunità che li accoglie a centinaia, per poter dare loro la possibilità di vivere. Ma tutto questo cosa può significare? Significa l'indifferentismo morale, lì evidentemente c'è il relativismo e, nella dimensione del relativismo, non c'è spazio nemmeno più per la dignità di ogni singola persona. Se c'è relativismo, inevitabilmente prevarrà il più forte sul più debole. E quindi noi ci troveremo che alcuni Stati e Governi riterranno di poter non dare una risposta a questo bisogno di aiuto e di non aprire le porte, che non significa evidentemente ancora una volta far entrare tutto e di tutto, dare il giusto sostegno. Ricordiamo l'ultima esperienza, quella dei corridoi umanitari, che hanno un fondamento di grandissima importanza: attraverso essi si dà la possibilità di arrivare in Europa, in quegli Stati dove si può assicurare una capacità di sopravvivenza, con la sicurezza e l'assistenza a livello non solo istituzionale, ma anche e soprattutto delle associazioni Grazie

trovato sulle sponde della Turchia. Ma ci sono migliaia e migliaia di Aylan, che non sono nemmeno approdati, da morti - lo devo dire

cui la guerra insistente, la povertà sfrenata e il terrorismo sono la causa principale della fuga di tanti innocenti (è così che li dobbiamo definire). Forse è tra tanti innocenti ci sarà qualcuno che vuole venire in Europa per altre delinquenziali azioni. In quel caso c'è bisogno di un' azione di *intelligence*, di un'azione di controllo, ma non si possono alzare muri e fili spinati in maniera generalizzata, perché nessuno possa entrare.

l'una, e lo voglio dire in maniera molto chiara e ferma: o l'Unione europea ha dei fondamenti di civiltà che sono stati definiti nella cultura giudaico-cristiana, oppure si è diventati così laicamente utilitaristici che, visto che

Non voglio fare polemica, ma alcune Regioni d'Italia, come la Lombardia e il Veneto, hanno buona possibilità di progresso economico proprio in ragione della presenza dei migranti.

«Mare nostro che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia, ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai da autunno per loro, da carezza, da abbraccio e bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

non so se la mia sarà una voce fuori dal coro, ma vorrei andare a monte e dire che c'è una cosa che a noi occidentali riesce proprio bene ormai da svariati secoli: ci arroghiamo il diritto di sapere cosa sia meglio per gli altri popoli del mondo.

Così partono le nostre missioni internazionali di pace, volte ad esportare la nostra poco disinteressata democrazia, creando odio e contrasti interni (l'altra faccia delle guerre civili), adducendo come scopo ultimo un mondo migliore per tutti. Grazie a questo metodo di azione nel 2015 sono morte nel Mediterraneo oltre 2.000 persone. Si tratta di gente costretta a fuggire dalla propria terra martoriata dalla guerra, rincorrendo la speranza di un futuro migliore per cercare un riparo. È così che donne, bambini e ragazzi rimangono vittime di annegamenti, protagonisti di una tratta di vite umane ridotte a mera merce di scambio. Per quanto tutto questo mi addolora, mi preme ancora di più sottolineare che non mi va di trincerarmi dietro un colpevole silenzio commemorativo della politica italiana, quella stessa politica complice della creazione di questa situazione. Più che di una giornata commemorativa c'è bisogno di agire, di dire le cose come stanno, fare nome e cognome dei colpevoli ed evitare il finto buonismo e il tentativo di generare una guerra tra poveri, tra cittadini e migranti. La responsabilità non può essere di chi fugge, ma di chi costringe a fuggire, ovvero di chi genera guerre devastanti nel nome degli interessi economici e delle speculazioni finanziarie, mascherandole come azioni di pace o di difesa dei nostri territori. Questo è ciò che è accaduto in Libia e sta accadendo anche in Siria. Le soluzioni che i tecnocrati di Bruxelles ci prospettano e che oggi sembrano andare per la maggiore sono la chiusura delle frontiere interne e lo scaricabarile verso quegli Stati più esposti, già martoriati a livello economico dalle politiche europee di austerità. Si vorrebbero abbandonare al proprio destino Stati come la Grecia e l'Italia e poi si fanno accordi con il signor Erdogan che viola in continuazione i diritti umani più basilari e minaccia di inondare i Paesi europei se non riceverà ciò che chiede: sostanzialmente distruggere indisturbato il popolo curdo. È così che si mettono in piedi missioni internazionali contro la Libia e poi si stringono accordi ed intese con l'Arabia Saudita che, nel 2015, ha fatto record di esecuzioni capitali tramite lapidazioni, impiccagioni e simili, per giunta in pubblico. D'altronde l'imperialismo che provoca l'immigrazione non può che trarre un profitto elevato dall'ingresso di nuove masse sfruttabili, per un gioco al ribasso basato sulla messa in competizione dei lavoratori migranti con i lavoratori italiani che genera una diminuzione di salari e diritti. Si investono molteplici risorse per gli armamenti, levando fondi utili per sanità, scuola e servizi sociali, per azioni militari imposte dalla NATO, e e quindi dagli Stati Uniti, verso quegli Stati da cui provengono i rifugiati per la gestione poi dei quali occorreranno altri fondi e quindi altro denaro. allora contro lo sfruttamento dell'immigrazione, ricordare le vittime di questo esodo, significa lottare contro quel sistema che dalla distruzione e ricostruzione di interi territori ci ricava bene e molto; lottare contro un sistema di accoglienza che non si occupa dell'effettiva protezione dei minori stranieri non accompagnati e che spariscono dai centri senza lasciare traccia per poi andare ad ingrossare le fila degli sfruttati da parte dei detentori del monopolio della delinquenza di strada. Per non parlare del meccanismo degli appalti dei servizi di accoglienza: Mafia Capitale insegna quanto ci si possa arricchire sulla pelle dei rifugiati a discapito poi dei poveri cittadini, che a malapena conservano qualche diritto sociale per loro stessi. Se non si è in grado di tutelare il diritto alla salute dei cittadini di questo Stato (e i dati odierni lo dimostrano) figuriamoci quello di coloro che sbarcano sulle nostre coste. Per questo dico che servono meno silenzi colpevoli in segno di rispetto e conseguenti giornate commemorative e più riflessioni sul fatto che i popoli devono conquistare il diritto ad una piena autodeterminazione e al controllo delle proprie risorse senza ingerenze esterne,

un tema importantissimo e, contrariamente ad uno dei colleghi che mi ha preceduto, ritengo sia assolutamente utile per creare consapevolezza di ciò che effettivamente è la migrazione e delle motivazioni che la determinano,

Ormai da decenni è in corso una vera e propria riscossa dei grandi poteri economici e finanziari e delle grandi *corporation* finalizzata a massimizzare i profitti passando sopra ai diritti umani, i diritti umani nei Paesi del cosiddetto terzo mondo e i diritti umani dei Paesi occidentali. La matrice è la stessa. La cosa che fa specie è che per motivi di convenienza politica

perché, se non la voteremo tutti, questo non sarà un esercizio ipocrita, ma sarà un esercizio di scelta politica, di appartenenza alla democrazia e ai valori della democrazia, dell'accoglienza, del rispetto verso le persone, della tutela dei diritti di appartenere a confessioni religiose, a etnie, a convinzioni politiche, ad orientamenti sessuali diversi.

cioè che era inutile, perché tutti siamo convinti del rispetto dell'altro e del fatto che l'altro che soffre e che fa una rappresentazione rappresentazione disperata della sua sofferenza trova in noi, tutti noi, quelle disponibilità che sono necessarie a chi soffre. Invece no, signor Presidente. Ci sono alcuni che dicono: «La sofferenza mi dà fastidio; vai a soffrire da un'altra parte, io non ti voglio vedere. Il dolore per me è raccapriccio, non voglio avere avere di fronte a me il dolore che tu rappresenti; risolviti i tuoi problemi da dove arrivi e, anche se non sei capace di risolverti quei problemi, la tua sofferenza tienitela a casa tua». Poi ci sono invece gli altri, quelli che hanno convinzioni diverse, democratiche, progressiste, aperte, che vivono nella relazione, che vorrebbero l'Italia e l'Europa terra di amicizia e di pace per i popoli; quelli che non vogliono i fili spinati, che sanno stare nella civiltà della globalizzazione, dove le relazioni sono imponenti ed importanti,

anche in questo Parlamento, rispetto alla nostra visione della cultura da mettere in campo, in relazione a questo e ad altri problemi.

i movimenti xenofobi, con vene profondamente razziste, antidemocratiche e irrazionali, anche sotto il profilo della relazione positiva sul piano economico e sociale. ci sono, crescono e fanno leva su paure che andrebbero invece eliminate, addirittura proposte per una riflessione di accantonamento e di superamento, tra individuo, società e comunità. Poi ci sono coloro che contrastano queste visioni. La tristezza politica, anche di questo Paese, è che coloro che pensano in termini democratici e progressisti - cioè coloro che pensano ad un futuro che non riporti l'Europa esattamente da dove viene, ovvero dalla parentesi devastante del nazionalsocialismo e del fascismo - si dividono attorno alle inezie, si dividono attorno alle inezie, a questioni particolari, specifiche e contingenti e non sanno ritrovare l'unità, che invece serve per far fronte a quelle spinte reazionarie, che arrivano ad essere sempre più consistenti, non solo nel nostro Paese, ma nell'intera Europa. Penso che proprio da questo provvedimento bisogna cominciare a capire se può esistere, in Europa e in Italia, una nuova dimensione culturale e politica, che metta insieme tutti coloro che pensano che la dignità umana e il valore della vita stanno sopra ogni cosa.

cercando di sfuggire alle tentazioni di discorsi importanti dal punto di vista valoriale e filosofico. Cercando di rimanere in questo ambito, dirò che stiamo per istituire una giornata della memoria, che è indirizzata, per quello che ci dice l'articolo 2, principalmente all'istruzione dei nostri giovani e quindi a sollecitare nelle scuole d'Italia un momento di riflessione e di attenzione ai fenomeni dell'immigrazione. Noi non possiamo non essere d'accordo su questo, ma a patto

di questi giorni ma tutta l'immigrazione e l'emigrazione che ha contraddistinto la storia del nostro Paese e in particolare della terra dalla quale provengo. Se nelle scuole della nazione siciliana si insegnasse la storia della Sicilia come storia del popolo siciliano, ogni capitolo conterrebbe una storia di immigrazione o di emigrazione,

si ricordi anche la nostra emigrazione che è immigrazione di italiani in altri Stati. Non è solo un fatto di reciprocità, ma proprio di educazione che noi dobbiamo dare ai nostri giovani. Molti studiosi hanno recentemente esplorato il fenomeno migratorio italiano, meridionale e siciliano in particolare, da e per le coste dell'Africa. La nostra

di cittadini (contadini, operai, commercianti, piccoli artigiani e anche imprenditori) recarsi in quella terra per portarvi la loro ansia di sviluppo, di crescita e di e di integrazione con gli abitanti di quella terra. Mi chiedo quindi perché, se non ci sono motivi - quelli sì

il disastro di Marcinelle o altri, cui abbiamo già dedicato una giornata di ricordo. Mi riferisco all'emigrazione che partiva con i piroscafi, senza sapere quale potesse essere la vera destinazione di chi disperatamente cercava di attraversare l'oceano, o all'emigrazione che sostava a Ellis Island. Peraltro, abbiamo visto anche recentemente una riscoperta dei valori e delle drammaticità attraverso importanti produzioni cinematografiche sulla storia dei nostri concittadini che emigrarono in passato. Di fronte all'idea di fossilizzare l'attenzione su un episodio drammatico, del quale naturalmente viene esaltata la data stabilendo che quello sarà il giorno della memoria, mi chiedo per così come noi chiediamo con gli emendamenti che abbiamo presentato e in base all'accoglimento o meno dei quali valuteremo l'atteggiamento da tenere in sede di votazione finale. Perché non andare nelle nostre scuole a parlare anche della nostra emigrazione, che ha toni altrettanto drammatici quanto quelli che oggi contraddistinguono la migrazione dall'Africa

ma perché limitare il discorso al Mediterraneo? L'emigrazione e l'immigrazione sono fatti epocali e storici che hanno contraddistinto gran parte dell'evoluzione sociale delle nostre popolazioni e, ripeto, in particolare della Sicilia, dalla quale provengo, per cui, molto spesso, noi, con un sorriso non dico sarcastico ma certamente di circostanza, ascoltiamo determinati discorsi che parlano di mura, che parlano di

che il contesto italiano e il contesto europeo ci assegnano come terra di frontiera, mentre noi siamo terra di centralità mediterranea. In base a questo, ripeto, chiediamo che il testo venga integrato da due semplicissimi emendamenti che sarebbero fondamentali e che e che mirano a far sì che nelle nostre scuole si parli non solo di immigrazione ma anche di emigrazione, in omaggio alla storia del nostro Paese, perché solamente questo omaggio potrà far comprendere meglio ai nostri giovani e alla nostra società i valori che, attraverso la giornata della memoria, si vogliono affermare. Non credo di

e al Governo di esaminare con attenzione l'opportunità di integrare il testo con i nostri emendamenti, ripeto che il nostro Gruppo Gruppo valuterà l'atteggiamento da assumere in dichiarazione di voto finale in base all'esito della discussione. E non mi si venga a dire che, siccome la Camera l'ha approvato, qui non si parla di urgenze. Tra l'altro, la Giornata della memoria è fissata il 3 ottobre, quindi c'è tutto il tempo, eventualmente, per un altro passaggio alla Camera, se si vuole iniziare da quest'anno a celebrare questa giornata. Non facciamo i soliti discorsi per i quali quest'Assemblea non è mai nelle condizioni di poter esprimere le proprie valutazioni e di poter esprimere un proprio voto diverso rispetto a ciò che accade o è accaduto nell'altro ramo del Parlamento, anche se siamo Si tratta di un disegno di legge assolutamente non impegnativo delle finanze pubbliche, né urgente per il nostro Paese, quindi credo che dovremmo affrontarlo con la massima serenità ed è per questo che chiedo vengano approvate le nostre proposte di integrazione.

Non affronterò le complesse questioni che il tema dalle migrazioni comporta, ma mi limiterò, invece, a prendere in esame ed affrontare la questione che oggi viene portata alla nostra valutazione attraverso questo disegno di legge,

La sollecitazione ad elaborare un disegno di legge che istituisse la Giornata nazionale della memoria per le vittime dell'immigrazione viene dal sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, e dal Comitato 3 ottobre, costituitosi appena alcuni giorni dopo il naufragio di quella data, che annoverava e tuttora annovera tra i suoi membri, tra gli altri, familiari e amici delle vittime di quel terribile naufragio. naufragio. Voglio entrare immediatamente nel merito di quella che risulta come la principale, ma forse la sola obiezione a questo disegno di legge: la principale, ma forse la sola perplessità che esso ha suscitato che possa trattarsi di un mero atto simbolico. Dico subito che un atto simbolico non è necessariamente superfluo. Un atto simbolico non è automaticamente inutile e tantomeno è destinato fatalmente a risultare dannoso. Nient'affatto. In questo caso, un atto simbolico può avere un suo significato molto denso e il motivo è semplice: gli atti simbolici, o meglio i simboli, i messaggi, le immagini, operano in un campo, abitano uno spazio, che è quello dove si formano le idee, dove si realizzano le opinioni, dove si costruisce il senso comune e dove si forma la mentalità condivisa. lì i simboli e gli atti simbolici possono acquisire una forza, una potenza che si traduce poi nel condizionare gli atti concreti delle persone, nel determinare gli orientamenti collettivi, nell'influenzare i comportamenti, i gesti dei singoli, dei gruppi e delle comunità. C'è, può esserci negli atti simbolici una forza e una materialità capaci davvero di indirizzare gli orientamenti collettivi. Dunque, un atto simbolico può avere questa potenza e ritengo che questo atto simbolico oggi sia ancora più necessario proprio perché, in materia di immigrazione e di asilo, assistiamo quotidianamente al ripetersi, all'intensificarsi sì di atti simbolici, ma di atti simbolici di ostilità, che producono diffidenza, che scavano fossati, che incentivano il conflitto etnico. Ebbene, da qui nasce la necessità di realizzare altri, diversi, positivi atti simbolici. Ecco, il contenuto profondo di questa iniziativa ‑ devo dire ‑ non ha alcuna intenzione polemica; non ha una volontà di contrapposizione, non vuole in alcun modo accentuare un dato che è obiettivo, ovvero quello della diffidenza da parte di alcuni strati della popolazione italiana, in particolare strati tra i più vulnerabili, più esposti, più deboli, nei confronti degli stranieri. Ha esattamente l'intento opposto: ha l'intento, cioè, di favorire l'incontro, di incentivare la relazione, il riconoscimento, la reciprocità, la riconciliazione. Tutto questo non è certo facile; non lo è in tutti i Paesi europei e in tanti sistemi democratici, ed è ancora meno facile, per certi versi, nel nostro Paese per una ragione che è già stata qui richiamata, richiamata, con intenti e accenti diversi, e persino con finalità diverse - ma che comunque penso siano tutti da valorizzare nell'intervento del senatore Micheloni, così come nell'intervento del senatore D'Alì, che pure sembrava andare in opposta direzione. il dato che io ritengo necessario evidenziare per spiegare la peculiarità di un atteggiamento della nostra società nazionale nei confronti dell'immigrazione? Penso che nella nostra società sia stata operata una grande rimozione, ed è esattamente la rimozione di quegli oltre 30 milioni di italiani che, come ricordavano i senatori Micheloni e Uras, dall'Unità d'Italia ad oggi sono partiti dal nostro Paese per cercare altrove, in altri Paesi e in altri continenti, un'opportunità di lavoro che era poi un'opportunità di vita e di futuro. Bene, questa realtà è stata come rimossa, ed è una realtà fatta di dolore, sacrificio, ma anche di conoscenza, di esperienza e di intelligenza. È stata certamente un'impresa travagliata, quella di quei milioni di italiani che hanno attraversato il mondo, ma è stato anche motivo di orgoglio,

Di questa straordinaria vicenda umana, che ha riguardato i nostri avi e nonni, in Italia si è quasi dispersa la memoria. Di questa straordinaria vicenda umana non si è fatta storia, non si è fatta narrazione, non si è fatta - passatemi il termine - epopea. devo usare intenzionalmente questo termine perché l'immigrazione poteva essere uno di quei miti fondativi della nostra identità nazionale che ha un'importanza notevole nel rafforzare il legame sociale, nel costruire identità e appartenenza. Ma questo non è stato fatto e quella vicenda umana è caduta nell'oblio. Della nave Sirio, di cui parlava il senatore Micheloni, che nel 1906 è affondata davanti alle coste spagnole con quasi 300 italiani finiti in fondo al mare e, più di recente,

non c'è memoria. Ma non c'è nemmeno memoria culturale, non c'è storia musicale, letteratura, né cinematografia di quelle vicende, perché di esse si è fatta, appunto, un'operazione di rimozione. E penso che proprio questa operazione di rimozione sia tra le cause principali dell'incapacità nostra - parlo proprio di noi tutti - di riconoscere nelle ansie, nelle speranze e nella sofferenza degli stranieri che arrivano in Italia l'ansia, le speranze e la sofferenza dei nostri avi e dei nostri nonni. E dietro c'è qualcosa che davvero va analizzato, ed è il fatto che un popolo come il nostro, che ha raggiunto nei decenni una qualche sicurezza economica, oggi messa a repentaglio dalla crisi ed erosa

perché richiama una povertà che si vuole lasciare alle spalle e di cui, in qualche misura, ci si vergogna. Ecco, il senso di una giornata della memoria sta esattamente qui: qui: nella capacità di creare una reciproca possibilità di riconoscimento tra tragedie che appartengono al passato, ma di cui dobbiamo conservare la memoria, e tragedie che sono dentro il nostro presente e che certamente sono destinate a durare nel tempo. E allora, davvero, non c'è nessuna retorica della solidarietà, non c'è nessuna enfasi del multiculturalismo in questo. C'è la necessità di

di far riconoscere l'altrui sofferenza non come un fatto pietistico, non come un atto compassionevole, ma come la sola base vera e reale di un agire politico. Non riesco infatti ad immaginare dove altro una politica all'altezza dei tempi possa trovare il suo fondamento, se non nella sofferenza degli esseri umani, nel loro bisogno di giustizia. Dove altro possiamo andare a cercare il fondamento del nostro agire politico? Certamente, l'Italia e l'Europa hanno bisogno di politiche intelligenti e razionali, che partano in primo luogo da un discorso che abbia a propria base demografia ed economia, ma tutto ciò non può fare a meno della consapevolezza di ciò che siamo stati e che altri popoli oggi sono. sono. La giornata della memoria può contribuire ad aiutarci in questa attività, certamente faticosa, perché la convivenza non è un pranzo di gala. La convivenza è qualcosa che può rilevarsi dolorosa, che può attivare conflitti e tensioni, ma è la sola alternativa al conflitto etnico. questa convivenza, che è il risultato di molta fatica e, temo, di molti dolori, è pero la sola via intelligente e razionale e, dunque, politica che, per me, può permetterci di affrontare fenomeni di tale portata storica e geografica con la giusta strumentazione. A tutto ciò, ovviamente, la giornata della memoria porta un contributo modesto, ma è appunto ciò che può aiutarci a far sì che quelli che chiamiamo troppo spesso, retoricamente, i nostri giovani, e che poi sono i nostri figli, non dimentichino di quanto dolore sia fatta la storia del nostro Paese.

denuncia resa pubblica nella giornata di oggi dalla Garante dei diritti delle persone detenute del comune di Bologna, che ha riportato il caso, in verità non unico nel nostro Paese, dato che riguarda decine di situazioni, di una donna rinchiusa nella casa circondariale della Dozza cinque e di diciotto mesi. Si tratta dell'annoso problema, che il nostro Paese non riesce a risolvere, della presenza all'interno delle carceri italiane di bambini, che stanno in carcere insieme alle loro mamme.

La legge n. 62 del 2011 prevedeva l'attivazione di strutture e istituti a custodia attenuata per le madri detenute

è stata messa in opera la rete delle case famiglia protette. Questa rete, la cui attivazione è stata affidata, dal punto di vista economico e dello sforzo finanziario, agli enti locali, fa una gran fatica ad essere attivata, perché un conto è una normale casa famiglia, altra cosa è una casa famiglia protetta che ospita madri detenute che devono scontare una pena (o che sono in attesa di giudizio, come nel caso di Bologna) con i loro bambini. Una casa famiglia protetta ha un costo molto elevato, motivo per cui, di fatto, gli enti locali fanno una gran fatica ad attivare

in ristrutturazione un'ala della sezione femminile del carcere di Bologna, che dovrebbe essere adibita a nido.

Nessun bambino deve rimanere all'interno delle strutture carcerarie nel nostro Paese e questo è un obiettivo che dobbiamo perseguire

sulla A19 Palermo-Catania. Ne sono crollati diversi, ponti e campate, e una risposta concreta a queste sollecitazioni ancora non c'è.

gli organismi preposti non si attivano. Cosa deve avvenire più di questo? Di cosa ci dobbiamo meravigliare? È tutto fermo e bloccato, ma perché? Non lo capisco e questo mi turba molto. Sono molto preoccupato anche per la nuova gestione, perché ancora non si capisce cosa sta programmando e avviando. Dal passato cosa esce? So solo che sono che sono entrati in campi sempre i soliti noti, i riciclati. Se dovete fare pulizia negli organi indicati, perché non cominciate a bastonare quelli che sono stati dentro questo sistema? Invece, forse vengono apprezzati. Se si viene riciclati nella politica è

voglio raccontare brevemente una storia di ordinaria follia, in cui la burocrazia vince su ogni ragionevolezza. Si tratta di uno strano caso che sta avvenendo in Abruzzo. È lo strano caso di Nelda Zazzara, una dipendente di scuola pubblica che ha versato per trentanove anni i contributi. Da circa un anno è molto malata e ha fatto, nel tempo giusto, la prima domanda di pensione per lavoratori "salvaguardati" (il 3 marzo 2014). La domanda viene accolta, ma la graduatoria scade. Le viene accolta la seconda domanda di salvaguardia il 4 dicembre 2014 (legge n. 147 del 2014), ma non accade nulla.

ma il Provveditorato agli studi si oppone e chiede, attraverso l'articolo 2 della legge n. 335 del 1995, l'accertamento dell'idoneità fisica, che si definisce con esito di non idoneità per sei mesi, fino al 15 In questo momento vengono parlate due lingue totalmente diverse; utilizzate due leggi diverse; ed è impossibile o, almeno, ogni tentativo è stato vano, far dialogare gli uffici. Per cui, da una parte c'è il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente, con la legge n. 274 del 1991, e dall'altra la non idoneità, peraltro temporanea, con la legge n. Sembra avvenire un ravvedimento quando l'INPS, a novembre 2015, comunica l'accoglimento della domanda di pensione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ma successivamente, con lettera del 19 febbraio 2016, l'INPS revoca l'accoglimento della domanda di pensione e avvia le procedure per il reinserimento lavorativo di Nelda, che nel frattempo, per ottemperare alle condizioni INPS, si era dimessa dal lavoro. Tutto ciò premesso, la signora Nelda, nonostante il riconoscimento di inabilità totale e permanente e circa trentanove anni di contributi, non riesce ad andare in pensione, ma non può nemmeno rientrare al lavoro, perché le hanno chiesto di dimettersi. Il caso è assurdo e rasenta la follia interpretativa e burocratica. Con un'interrogazione chiedo al ministro Poletti di intervenire sugli uffici competenti e sull'INPS, perché si ridia, con equilibrio e senso di giustizia, senso a questa vicenda, richiamando gli uffici che hanno sbagliato, sicuramente la ragioneria del Provveditorato, o quali altri organi si siano erroneamente espressi, e trovando la soluzione più rapida, giusta e anche meno onerosa per lo Stato.